Onorevoli colleghi, sull'incidente avvenuto ieri in una fabbrica di Arpino ha chiesto di intervenire il Presidente della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, al quale do subito la parola.

ringrazio, signora Presidente, per l'attenzione che il Senato vuole rivolgere ad un fatto così drammatico che ritengo abbia scosso la coscienza di tutti i cittadini italiani. La ringrazio inoltre per aver voluto onorare non solo e soltanto i lavoratori che sono morti ieri durante lo svolgimento della propria attività,

nel comune di Arpino, in località Carnello, ha fatto nascere in noi tutti sentimenti vari di cordoglio, di sgomento, di dolore, di disperazione, di solidarietà, di vicinanza nei confronti delle famiglie. È morto il titolare dell'azienda, con due figli, oltre ad altri due lavoratori ad una persona, un avventore che si ritiene che in quel momento si trovasse sul posto. Vi sono state due esplosioni, due enormi deflagrazioni che hanno distrutto tutto. Allora, viene alla memoria che questo è un settore che va maggiormente attenzionato, se è vero, come è vero, che nella provincia di Frosinone, negli ultimi 22 anni, vi sono stati ben cinque episodi di questo tipo, con 19 vittime.

Sono dati che debbono farci riflettere, che debbono porci nelle condizioni di attenzionare ancor di più questo settore, e di comprendere cosa si può e si deve fare per evitare che vi siano, stando ai numeri che ho detto, percentuali che vanno al di sopra di ogni altra tipologia di lavoro, in riferimento al rischio e alle vittime. Questo noi non lo possiamo più permettere. Domani, alle ore 14,30, è stata già convocata la Commissione che si interessa, appunto, di questi gravi temi della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Io desidero ringraziare ancora una volta il presidente Schifani, che ha avuto la sensibilità di voler

cercando di porre all'attenzione una serie di problematiche che ancora esistono e che hanno bisogno di risposte. Io mi auguro che questa tragedia,

delle condizioni del lavoro delle fabbriche di fuochi artificiali, perché non si ripeta quanto, purtroppo, spesso si determina. Noi faremo del nostro meglio, signora Presidente, e vogliamo ritenere che, al più presto, avremo elementi maggiori da poter riferire all'Aula. Nel momento in cui andremo con una delegazione sui luoghi, apriremo formalmente e ufficialmente la nostra inchiesta, per far sì che anche quest'Assemblea, che ha voluto un'importante Commissione in un settore così delicato, possa avere maggiori elementi e maggiori dettagli. Mi permetto di concludere, signora Presidente, pensando ancora alle parole che il Presidente il Presidente della Repubblica ieri ha voluto rivolgere alle famiglie, ma anche a tutta l'Italia e a tutti gli italiani in un momento così difficile e delicato.

intendo anch'io esprimere il più profondo cordoglio, mio personale e del Gruppo del PD, alle famiglie delle vittime e alla comunità locale per la gravissima esplosione che si è verificata ieri ad Arpino in provincia di Frosinone, dove hanno perso la vita, a seguito di un grave incidente in una fabbrica di fuochi d'artificio, sei persone: i titolari dell'azienda, due operai e un addetto di un'altra società del settore. Si tratta di una vera e propria nuova strage sul lavoro, una delle più gravi avvenute negli ultimi anni in Italia. Ancora una volta l'incidente riguarda una fabbrica che tratta materiali ad alta pericolosità come i fuochi d'artificio: un settore ad alto rischio dove la prevenzione e le prassi devono essere certificate con la massima attenzione. ripropone drammaticamente il tema degli incidenti sul lavoro, una piaga che in Italia continua ad essere spaventosa: nel solo 2011 si registrano più di 350 morti. Ed è bene ribadire, ancora una volta in quest'Aula, che sento un po' indifferente, che la crisi economica non può in alcun modo rappresentare una giustificazione per allentare controlli ed ispezioni. Non servono le ispezioni a tragedia avvenuta: invece assumere più ispettori, e serve non emanare circolari che, come avvenuto in passato, allentino le ispezioni; serve non fare leggi, come l'articolo 8 della manovra economica, che indeboliscono fino ad annullare le normative nazionali; soprattutto, servirebbe coinvolgere la piccolissima impresa in processi di formazione, e far comprendere che una norma in più non salva la vita solo ai lavoratori, ma anche ai piccoli imprenditori. Servono corsi di formazione seri e verificati, sanzioni efficaci per i titolari delle fabbriche e delle aziende che non rispettano le norme di sicurezza. È indispensabile che, accanto al lavoro di indagine della magistratura e di ispezione dei servizi ministeriali già annunciati dal ministro Sacconi, a cui chiediamo di riferire quanto prima in quest'Aula sull'accaduto, le istituzioni e le parti sociali si attivino per comprendere meglio qual era il livello di procedura organizzativa applicato nelle lavorazioni in base alla documentazione dei rischi, il livello di formazione e preparazione degli addetti, la qualità dei materiali. Ciò al fine di attivare misure concrete capaci di non farci più assistere a tragedie di tale portata. Mi associo alle parole del presidente Tofani e al lavoro che la Commissione sta svolgendo in maniera unitaria.

che quando un uomo, una donna o un ragazzo muoiono per il lavoro, il problema dovrebbe toccarci come prima questione del nostro operare nelle istituzioni. E infine, vorrei ricordare

Signora Presidente, il Gruppo della Lega Nord si unisce alle parole di cordoglio espresse in quest'Aula dai Gruppi politici presenti. Purtroppo, dobbiamo constatare ancora una volta come, davanti a tragedie e a morti sui luoghi di lavoro, le cosiddette morti bianche, si spendano forse troppe parole senza essere esattamente a conoscenza di

in tante altre parti del Paese. Sarà la carenza di personale, sarà forse la mancanza di volontà da parte di qualcuno, ma questa è la realtà. Dobbiamo continuare nel nostro lavoro di favorire

nell'azienda «Pirotecnica Arpinate». La tragedia avvenuta ieri in Provincia di Frosinone è solo l'ultimo dei tanti drammatici episodi che registriamo continuamente. Le vittime del lavoro sono state solo nel 2011 La media è di tre morti al giorno. La sicurezza sul lavoro, come ha già sottolineato oggi anche la CGIL, è ancora una grave emergenza. Tanti incidenti riguardano i lavoratori extracomunitari assunti in nero, che rappresentano ben il 40 per cento dei morti sul lavoro, e non è un caso che ogni tanto si abbia notizia del ritrovamento sul ciglio della strada, a pochi passi dai cantieri, di qualche cadavere. Ma torniamo alla tragedia di ieri. Essa dimostra che senza un rafforzamento dì controlli certi, finalizzati alla prevenzione degli incidenti, in particolare nei settori più a rischio, le morti sul lavoro continueranno ad aumentare. Sono necessari maggiori controlli, specialmente in siti ad alto rischio, come era quello di Arpino. Sul suo *blog* ieri il ministro Sacconi ha scritto che «i servizi ispettivi del Ministero del lavoro sono stati già attivati affinché collaborino con i Vigili del fuoco, con il Servizio sanitario regionale e con gli inquirenti al fine di una tempestiva individuazione delle cause e delle eventuali responsabilità». Ma ciò non basta. Non si può intervenire solo a tragedie avvenute. Lo sbandierato Piano triennale del lavoro presentato dal Governo quasi un anno fa avrebbe dovuto vertere sulla lotta al lavoro irregolare e sull'aumento della sicurezza sul lavoro. Finora si sono indicate non meglio definite «azioni di vigilanza selettiva» e «modifiche ai sistemi sanzionatori che ne accrescano l'efficacia». Come abbiamo già avuto modo di dire più volte, anziché «lotta al lavoro irregolare» si sarebbe dovuto più brevemente e correttamente scrivere «lotta alla sicurezza sul lavoro», visto che dall'inizio della legislatura il Governo si è applicato con costanza solo al sostanziale smantellamento delle tutele previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Ulteriori modifiche in senso peggiorativo sono peraltro previste dal cosiddetto disegno di legge di "semplificazione", per fortuna - e speriamo mai lo sarà - non approvato. il Governo, anche con l'ultima manovra, ha attuato solo tagli nelle attività ispettive e di controllo, provocando un rallentamento delle ispezioni, ormai evidente. La manovra peggiorerà sicuramente la situazione. Mentre si discute molto di auto blu, gli ispettori della sicurezza devono molto spesso usare mezzi propri e senza avere il carburante necessario. Signora Presidente,tutto questo è davvero inaccettabile. Impegniamoci di più per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro a tutti i lavoratori.

il cui appello va raccolto - a proposito di un settore che di per sé manifesta una pericolosità di fatto e che dunque induce all'esigenza di un accompagnamento e di un'attenzione ancora più forte rispetto ad altri settori, ma anche perché la tragedia che abbiamo di fronte è la tragedia del lavoro tutto intero, di chi fa l'imprenditore e di chi fa il lavoratore. In quella tragedia è morto il padrone ed è morto il lavoratore: sono morti tutti quelli che in un'«azienda comunità», qual è la piccola azienda, lavorano e contribuiscono all'impresa, al di là

manifestano un continuismo ideologico che qualche volta dovrebbe fare i conti con la realtà e aiutarci ad avere un senso di pietà, senso di pietà, di ragionevolezza e di comprensione, che forse aiuterebbe tutti noi a fare meglio il nostro lavoro, oltre che ad esprimere il cordoglio, con convinzione e consapevolezza.

un recente taglio economico ad aver prodotto questi numeri così elevati, che perdurano da troppo tempo, anche in relazione

personale cordoglio e quello dei senatori del Gruppo Per il Terzo Polo alle famiglie delle vittime per il terribile incidente di Carnello di Arpino, nel frusinate. un cordoglio vero e sincero, perché sono morti il proprietario dell'azienda e i figli, gente che da sempre lavorava in quel settore, un settore particolare, molto difficile e molto pericoloso.

e sincero cordoglio per quella famiglia. In questi anni, insieme al presidente Tofani - che vorrei ringraziare - e insieme a tutti gli altri componenti della Commissione

che, benché in Italia ci sia un numero doppio o triplo di operatori che controllano e lavorano nel campo della sicurezza sul lavoro, il numero dei morti che verifichiamo in Italia è doppio o triplo rispetto a quello delle Nazioni più moderne d'Europa. Questo ci deve spingere a una grande riflessione e a pensare che probabilmente va rivisto tutto il sistema dei controlli,

i proprietari, coloro che tutti i giorni vivono l'azienda, perire in un gravissimo incidente. L'altra settimana nella mia città, ad Anzio, si è verificato un altro gravissimo incidente,

che però noi viviamo e soffriamo in questo momento, dobbiamo rivedere secondo me tutta la filosofia della sicurezza sul lavoro, partendo dalla prevenzione e passando anche ai discorsi sanzionatori, rivedendo tutto ciò che riguarda la sicurezza in Italia, perché di lavoro si deve vivere, ma non si può morire.

Signora Presidente, colleghi senatori, ad integrazione e completamento della relazione scritta desidero fornire alcuni ulteriori elementi

e a legittimare, per altro verso, la richiesta di una valutazione positiva da parte dell'Assemblea. Nella prima stesura, quella originaria, la proposta di legge faceva riferimento esclusivamente a due enti, ai a due enti, ai quali veniva affidato il compito di promuovere la ricerca nell'ambito di quella cultura e di quella storia latina e medievale

a quell'immaginario dei castelli e delle cattedrali che in qualche maniera ciascuno di noi porta nel proprio vissuto e nella propria cultura individuale. I due enti erano il SISMEL (Società internazionale per lo studio del medioevo latino), con un finanziamento iniziale di 1.500.000 euro, e l'ENTMI (Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia), con 500.000 euro. Nel corso dei lavori presso la VII Commissione della Camera, l'onorevole Manuela Ghizzoni del Partito Democratico, dopo aver evidenziato e sottolineato la positività e l'urgenza dell'intervento dell'intervento legislativo, rimarcava però come mancassero a suo avviso altri enti ugualmente meritevoli di attenzione, e citava in particolare l'Istituto storico italiano per il medio evo e il Centro italiano di studi sull'alto medioevo di Spoleto. All'unanimità veniva quindi scelto il percorso dell'attivazione di un Comitato ristretto che doveva appunto arrivare nelle intenzioni dei commissari ad una stesura unitaria. Con due successive riunioni - quindici minuti in tutto, a indicare che non vi sono state particolari problematiche - si arrivava a una formulazione condivisa all'unanimità: quella che sostanzialmente ci troviamo ad esaminare oggi in questa sede. Il documento, con l'approvazione della Commissione (che aveva chiesto addirittura il trasferimento in sede legislativa, a testimonianza del fatto che vi era un'assoluta convergenza delle posizioni), passava quindi all'Assemblea, dove in tutte le votazioni intermedie si registrava un consenso particolarmente ampio. I primi quattro articoli, che sono poi il cuore del provvedimento, venivano approvati con un solo voto di astensione. In sede di votazione finale, su 485 presenti, vi sono stati solo quattro contrari e 190 astenuti, come emerge dalle dichiarazioni di voto, che hanno sottolineato, per un verso la positività del provvedimento, e quindi

Ho voluto brevemente ripercorrere questi passaggi perché in qualche maniera rendono conto della convergenza da parte di tutte le forze politiche sull'utilità di quel provvedimento, in maniera assolutamente trasversale, perché, al di là di tutto, si vanno a finanziare degli enti assolutamente meritori, seppure in un ambito limitato, definito e ristretto. L'alternativa sarebbe quella di rinviare tutto, di fermare questi finanziamenti, che hanno trovato peraltro una loro legittima copertura. Quindi, il rischio è eventualmente in questa direzione. Non nascondo, nella mia veste di relatore (peraltro queste riflessioni compaiono nel documento accompagnatorio a mia firma), la sostanziale anomalia del ricorso allo strumento normativo primario per una finalità di questo genere. Quindi, tale procedura denota in effetti elementi che possono destare destare perplessità e dei momenti anche di incertezza; però, a mio giudizio deve in qualche modo prevalere il buon senso: alla forma bisogna sostituire la sostanza, e la sostanza è quella di un'iniziativa necessaria, che viene definita importante da tutte le parti politiche. Obiettivamente, rinunciare a questa opportunità sarebbe un atto assolutamente privo di responsabilità.

tuttavia, pur di non perdere almeno le risorse residue, ci accingiamo a dire perché ci stanno a cuore anche questi istituti. I quattro istituti, come gli altri, hanno necessità di essere sostenuti anche per valorizzare un tempo della nostra storia e della civilizzazione occidentale. I non studiosi dell'Evo Medio hanno reminiscenze di carattere scolastico o evocazioni letterarie, spesso segnate da giudizi approssimativi e non corretti. L'espressione della *vulgata* corrente è che si è trattato di secoli bui. Secoli sì, perché fu un periodo molto lungo, ma

È stato un periodo che amerei definire luminoso, per l'irradiazione delle culture dall'Italia al Centro e al Nord Europa: la filosofia, la pittura, la lingua. Le lingue neolatine da lì hanno trovato origine e radice. Un lungo tempo che non ha disprezzato né disperso il passato ed ha preparato il futuro. Non ha cancellato neppure le feste e, con una sapiente azione di integrazione culturale, ha cristianizzato celebrazioni precristiane e pagane, convertendole.

Dalla latinità alla cristianità l'Europa ha integrato differenze di ordinamenti giuridici, di scambi economici: conoscere il Medioevo significa ridare radici al nostro oggi. *(Brusìo).* Ridare radici al nostro oggi vale anche per chi coltiva, difende e aggiorna la nostra lingua. È noto, e si sentirà in quest'Aula, il rimpianto

Basta poco, anche ad osservatori non specialisti, per accorgersi di quanto la nostra lingua abbia necessità vitale di essere difesa e fatta conoscere, e questa è la missione dell'Accademia. Una lingua povera, meticciata, strapazzata rovinata da un lessico da strada lede la tradizione stessa del sapere del nostro Paese. Questo Governo, dal primo atto di rilievo - la manovra estiva del 2008 - ha dimostrato con i fatti quanto poco abbia a cuore la cultura del nostro Paese e la transizione e la tradizione di una grande cultura alle nuove generazioni. Senza lingua si è senza pensiero, si è senza anima. Non basta ascoltare un po' in giro i discorsi per capire a che livello qualitativo è stata ridotta la lingua italiana. Quanti sono i vocaboli che vengono usati? C'è un impoverimento incredibile. Qual è la comprensione del significato della lingua italiana da parte di chi legge i giornali o un libro? Abbiamo davvero bisogno che una cultura linguistica garantita dall'Accademia della Crusca possa vivere. Pertanto il nostro pensiero sulla politica culturale del Governo non può cambiare, a meno che non cambi la politica e, con rammarico, ci troviamo ad operare una scelta incresciosa:

Se lo spirito e la pacatezza con cui ricordiamo quanto deve stare a cuore al Parlamento italiano, che guida il presente ed il futuro del Paese, il dibattito al quale ci siamo accinti, probabilmente possiamo chiedere ai colleghi di votare a favore degli emendamenti Nel caso in cui questo ripensamento avvenga - e sarebbe atto meritorio del Senato - è di tutta evidenza che cambierebbe anche il nostro atteggiamento e il giudizio che mi sono permessa di esprimere (anche se sarebbe dovuto essere invece un giudizio pesante ed urlato) nel richiamare la necessità di una politica culturale che diventi priorità.

noto innanzi tutto con piacere che questo disegno di legge riunisce esponenti di forze politiche differenti, alcune di maggioranza,

Probabilmente, la scelta del disegno di legge è servita anche a superare alcune resistenze governative e a consentire al Parlamento di recuperare una sua centralità, dando impulso ad un investimento nella cultura che in questi anni purtroppo non si è avuto. Esso appare quindi in controtendenza rispetto ad una politica che ha visto pesanti definanziamenti nei confronti della cultura in generale e in particolare nei confronti degli istituti che ora invece ottengono alcuni nuovi finanziamenti.

Vi è poi un altro aspetto che depone a favore di questo disegno di legge, vale a dire l'oggetto specifico, il finanziamento di istituti e di fondazioni che si occupano del Medioevo; un'epoca storica fondamentale per la costruzione della nostra identità nazionale. È nel Medioevo che nasce la lingua italiana. È nel Medioevo che si inizia a modellare l'identità italiana e che si definisce l'identità europea. Il Medioevo è anche un'epoca di straordinaria attualità, perché si fondono popoli diversi, si sviluppa una cultura unitaria all'insegna di quell'incontro-scontro, che tuttavia diventa fecondo ed estremamente positivo,

Probabilmente bisognerebbe inserire simili iniziative in una più ampia revisione della disciplina che

la necessità di una selezione dei finanziamenti in senso fortemente meritocratico per individuare le punte di eccellenza ed evitare una dispersione di finanziamenti. pertanto al Governo di avviare una revisione generale della disciplina della contribuzione e approfitto di questa occasione, sicuramente felice, per lanciare un appello al Ministro della cultura e al Governo in generale. Con riferimento alla opportunità di finanziare... *(Brusìo).* PRESIDENTE. Colleghi, non posso davvero consentire che il senatore Valditara debba urlare per farsi sentire.

proprio in virtù della finalità che ho cercato di sottolineare all'inizio di questo mio breve intervento, cioè quella di valorizzare lo studio delle radici della identità italiana, come non immaginare di estendere questi finanziamenti anche ad altri istituti, ad esempio all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo, ad esempio alle unità di ricerca del CNR

fare un discorso di carattere più generale proprio per tracciare un percorso che arrivi sino ad oggi, passando ovviamente per il nostro Risorgimento, da Roma al Medioevo, sino all'Ottocento, proprio

un piccolo cambiamento di rotta in cui il Parlamento diventa protagonista, e quindi certamente il nostro Gruppo parlamentare voterà a favore, e coglie questa opportunità anche per lanciare un segnale affinché questo tipo di iniziative non siano dei

vorrei spiegare il nostro atteggiamento di non piena condivisione del provvedimento al nostro esame. Vorrei dire subito con grande chiarezza che non è per il merito,

Le nostre domande, che riproponiamo oggi al Governo - se il senatore Gasparri mi consente e consente al sottosegretario Villari di ascoltare, se vuole, l'intervento, anche perché sto appunto parlando di domande che abbiamo posto al Governo nella discussione in Commissione e che riproponiamo in in questa sede - riguardano i criteri adottati per approvare una legge che sostiene soltanto alcuni istituti (quattro per la precisione) con più di due milioni di euro, vale a dire quasi un terzo dello stanziamento complessivo a favore degli istituti culturali, che è stato, com'è noto, dimezzato nel 2010, mentre ad altri si tagliano risorse. Sono istituti sicuramente importanti quelli oggetto di questo provvedimento, che meritano di essere sostenuti, ma non sono certo gli unici a trovarsi in ristrettezze economiche. Abbiamo chiesto al Governo che cosa si prevede per il futuro delle altre istituzioni che rientrano nella tabella della legge n. 534 del 1996, che cosa il Governo intende fare per altre istituzioni prestigiose che versano in grandi difficoltà fino a rischiare di chiudere per mancanza di risorse sufficienti. Porto ad esempio l'Accademia della Crusca (la senatrice Garavaglia lo ha già fatto) perché questa è particolarmente significativa, ma potrei citarne altre ugualmente prestigiose, lasciate in agonia. La Crusca non ha ancora chiuso i battenti (bisogna che i colleghi ed il Governo questo lo sappiano) semplicemente perché la Regione Toscana l'ha finora sostenuta e anche per questa istituzione, fra l'altro, c'è una proposta di legge e sarebbe stato un modo intelligente di celebrare il 150° dell'Unità d'Italia finanziare il massimo organismo preposto allo studio, alla ricerca storica e alla promozione della nostra lingua nel mondo. E invece niente. Tutto è fermo. Solo promesse. Anche gli impegni assunti in 7a Commissione attraverso l'approvazione con voto unanime - lo sottolineo - di un ordine del giorno che prevedeva uno stanziamento congruo di risorse a suo favore come a favore degli altri istituti, sono stati disattesi. Rigettando i nostri emendamenti, il Governo, con poche e scarne parole ha motivato il suo no con una non idonea copertura finanziaria. Ma è chiaro a tutti che non è la copertura il problema. Se ha la volontà politica di sostenere istituzioni culturali di grande prestigio e utilità, il Governo trovi una copertura più adeguata. Ma esca dall'imbarazzo e dal penoso balbettio che l'ha caratterizzato finora. Vorrà dire qualcosa se anche il relatore ha espresso perplessità. Per noi è davvero poco comprensibile soprattutto se mettiamo in fila, signora Presidente, colleghi, i ripetuti tagli di cui la cultura è stata oggetto durante tutto l'arco di governo del centrodestra. La risposta del Governo alle nostre sollecitazioni in varie occasioni è stato - com'è a tutti noto - l'azzeramento dei contributi in una prima versione della manovra di maggio e poi addirittura la soppressione di enti e istituzioni importanti nell'ultima manovra in via di approvazione alla Camera. Faceva una certa impressione leggere nel cosiddetto decreto sviluppo di maggio che a decreto approvato «lo Stato cessa di concorrere al finanziamento degli enti, istituti, fondazioni e altri organismi», indicati in un elenco allegato: 232 istituti che avrebbero dovuto arrangiarsi da soli a prescindere dalla loro attività e validità. approvato dal Governo addirittura si è pensato bene di tagliare la testa al toro e di sopprimerne del tutto alcuni. In entrambi i casi per fortuna - grazie all'intervento del Capo dello Stato e alla pressione dell'opinione pubblica il Governo è stato costretto a una marcia indietro, per quanto parziale nel primo caso: il contributo è stato infatti soltanto dimezzato. Resta il fatto che questo Governo ha provato in tutti i modi a chiudere i rubinetti alla cultura, anche teorizzandolo con le famigerate parole del ministro Tremonti: con la cultura non si mangia. Visione miope e meschina di un Paese, di un popolo, direi di una Nazione che si identifica anche e soprattutto per la sua cultura, per la sua storia, per la sua tradizione. Aggiungerei: una visione povera della democrazia che porta a scelte di corto respiro che rientrano in una visione della politica economica che non investe sullo sviluppo e sulla crescita, ma si limita a contenere la spesa e a tagliare risorse anche in settori cruciali come la formazione, la ricerca, l'innovazione: il sapere e la cultura, appunto. Si pensa di poter abbandonare interi settori culturali al mercato, di affidarli al privato. Ma è evidente che così non può essere. La cultura ha bisogno prioritariamente dell'investimento pubblico. Come viene documentato da un recente rapporto di Federculture, infatti, gli investimenti privati si riducono se si riducono quelli statali, soprattutto in assenza di politiche fiscali che rendano conveniente per le imprese e per i cittadini investire in cultura. È dunque un tessuto ricco e importante che si sta lacerando. Ma perché tanto accanimento verso istituzioni senza scopo di lucro, che promuovono attività di studio e di ricerca, che mettono a disposizione della pubblica fruizione preziosissimi patrimoni librari e archivistici, che sono tra i soggetti più attivi nel campo della pubblicazione di volumi e di prodotti editoriali, che promuovono borse di studio per giovani studiosi e organizzano attività formative e di aggiornamento, offrono straordinarie opportunità di crescita civile e culturale, che svolgono un servizio pubblico in sostituzione dello Stato e sono spesso un modello significativo di sussidiarietà tra privato e pubblico? Queste istituzioni sono infatti spesso delle vere e proprie eccellenze - tutti lo devono sapere - che gestiscono patrimoni privati, ma che appartengono alla storia collettiva del nostro Paese, e non possono essere disperse, pena la perdita della nostra memoria storica e politica. Fanno parte di quel valore cultura che, se adeguatamente considerato e promosso, potrebbe aiutare a realizzare la crescita economica, oltre che civile e sociale, del nostro Paese. Non è retorica. Così ha fatto e continua a fare, anche per uscire dalla crisi economica, la Germania, Germania, come anche la Francia. Non a caso, uno dei più autorevoli settimanali tedeschi, «Die Zeit», nel luglio scorso ha dedicato un'edizione all'elogio della cultura nella quale si metteva in risalto l'enorme offerta culturale della Germania, considerata la misura della civiltà di quel Paese. In Italia si preferisce invece deprimere tutto ciò che produce e promuove cultura, considerata un peso insostenibile. Noi non ci arrenderemo e proseguiremo con le nostre e proseguiremo con le nostre denunce e con le nostre proposte convinti - come Martha Nussbaum nel suo «Non per profitto» - che se si continueranno ad espungere quei saperi che «sono indispensabili a mantenere viva la democrazia, i Paesi ben presto produrranno generazioni di docili macchine anziché cittadini in grado di pensare da sé, criticare la tradizione e comprendere il significato delle sofferenze e delle esigenze delle altre persone». Saranno democrazie forse senz'anima, se possibile, prive di civiltà, di coesione, di capacità di riconoscimento reciproco. Ed allora, anche per impedire che si diventi tutti delle «docili macchine», vogliamo che si mantenga la ricchezza culturale rappresentata e coltivata anche dai molti enti di eccellenza ben noti al pubblico.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, è mio parere che si debba accogliere con favore la direzione in cui si muove questo provvedimento e anche la sostanza dello stesso. La prima ragione è che si interviene a sostegno degli studi relativi ad una grande epoca di radicamento della nostra storia e della nostra identità, che ha sofferto più di altre in passato. I colleghi debbono infatti avere memoria, sia per avere avuto esperienza dell'argomento in più legislature, sia per essersi occupati della materia, che è un settore che ha sofferto più di altri della decurtazione di risorse e delle strumentazioni e delle indagini della ricerca. È comunque un tempo della nostra storia e della nostra identità che, a livello italiano ed europeo, merita il massimo dell'impegno, dell'approfondimento e della divulgazione. La seconda considerazione è che effettivamente mi sembra si intervenga nei confronti di istituti che esprimono il massimo della capacità di produzione culturale e della ricerca.

il Centro italiano di studi sull'alto medioevo fu, in particolare, voluto dal magnifico rettore dell'università degli studi di Perugia, senatore e professore Giuseppe Ermini, che è stato un grandissimo promotore della cultura e, in particolare, degli studi storici a livello italiano ed europeo, oltre che promotore di convegni di grandissimo lignaggio.

non è trascurabile. Si tratta quindi di un intervento non meramente simbolico. Certo, ci sono altri istituti che, sia pure in altri settori, con approfondimenti verso altre epoche e aspetti della nostra storia identitaria, meriterebbero sostegno, ma i tempi sono quelli che sono. D'altra parte, una frammentazione estrema, spinta fino all'eccesso, delle risorse, porta come conseguenza che dare una briciola ciascuno significa non dar nulla ad alcuno. Significa intervenire in maniera assolutamente impercettibile e priva di qualunque risultato pratico. Infine, vorrei dire, è abbastanza importante sul piano politico che ci sia stato un incontro di volontà tra l'iniziativa parlamentare di vari colleghi di diversi Gruppi e il consenso concreto del Governo, che ha dimostrato, pur nelle ristrettezze presenti, una sensibilità culturale ed una volontà, sia pure in misura non adeguata e certamente insufficiente, rispetto alle aspirazioni e alle aspettative di venire incontro a quelle istanze. Non mi sembra affatto un'anomalia che ci sia stato l'incontro virtuoso di volontà tra il Governo e i proponenti di livello parlamentare. Magari - starei per dire - ci fosse in tanti altri campi e in altre materie un tipo di incontro

proprio a quegli studi, che non sono astratti, remoti, non sono esercitazioni accademiche, ma sono la riscoperta dei fondamenti, delle ascendenze precise di ciò che siamo culturalmente e di ciò che possiamo continuare ad essere in Italia, in Europa e nel mondo. Quindi, auspico

In primo luogo, non mi pare giusto e corretto mettere in contrapposizione gli enti di cui ci stiamo occupando con altri prestigiosi, anche se in ambiti diversi. Il testo reca «Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo», per cui a questi enti dobbiamo in qualche modo riservare e limitare l'attenzione. È stato detto da più parti che con la cultura si mangia. Mi sia consentito dire che mai mi sono trovato più d'accordo con una tesi sostenuta dalla sinistra. Sono testimone che per decenni

della mia provincia. Centinaia di persone inefficienti sulla cultura hanno costruito patrimoni. È quindi vero che con la cultura si mangia, ma non si dovrebbe mangiare in detto modo. Dico questo per chiarire che, se oggi viviamo momenti difficili, è proprio perché alle spalle abbiamo esperienze tutt'altro che positive. dalla senatrice Franco, ho già presentato le mie valutazioni e ho sottolineato come lo strumento normativo primario sia, a mio giudizio, anomalo e inopportuno. Si tratta in questo caso, però, di valutare se, al di là del metodo, che sicuramente può trovare valutazioni anche di censura, dobbiamo salvare il merito del provvedimento, e comunque tener conto che vi sono due milioni di euro a disposizione di enti

è stato ricostruito, dal relatore e dagli interventi che mi hanno preceduto, l'*iter* di questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che reca la concessione di contributi a quattro enti che svolgono ricerca sul Medioevo, un'epoca oscura. In un primo tempo, si era indirizzati a sostenere una platea ancora più ristretta di enti e istituti che approfondissero quell'epoca della nostra storia e della storia europea. Tengo a sottolineare che questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare arriva qui al Senato dopo che alla Camera tutte le forze politiche in Commissione, come bene ha ricordato il relatore, hanno individuato i quattro enti che affrontassero in maniera organica le tematiche connesse a questa opera. È difficile oggi, come abbiamo detto nel lavoro e nel confronto in Commissione al Senato, contrapporre enti e istituti tutti, meritevoli di sostegno. Precedentemente al precipitare della crisi congiunturale internazionale, in ogni caso, si sono riusciti a recuperare risorse per sostenere e stabilizzare quanto è nelle nelle prerogative degli enti individuati. Certamente rammarica tutti noi il fatto che istituzioni prestigiose, che sono già state citate e che io non citerò di nuovo, meritassero ugualmente il sostegno. Il criterio e la modalità che il Governo ha adottato, nel rispetto del lavoro parlamentare, di accompagnare questo disegno di legge con la copertura richiesta che, in qualche mondo, era condivisa e ha raggiunto una sostanziale unanimità nel passaggio alla Camera.

che qui riporterò brevemente, la cultura è il settore che concorre al PIL europeo in maniera più rilevante. La cultura in senso lato incide per il 5 per cento sul nostro PIL. Ogni euro investito in cultura ne genera poco meno di tre. Ogni posto di lavoro promosso in questo comparto ne richiama nell'indotto poco meno di altri due. Quindi, la cultura è un grande volano di sviluppo che, accanto a quelli che sono che sono beni immateriali, concorre a riscoprire l'identità del nostro Paese; che, in qualche modo, rilancia la nostra storia e la nostra tradizione che, grazie a Dio, non sono replicabili da altri

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, il parere è di nulla osta ad eccezione che sull'emendamento 3.0.203 sul quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «per il triennio 2011-2013» con le seguenti: «per il biennio 2012-2013». In relazione, poi, agli emendamenti 3.0.200, 3.0.201 e 3.0.203 (ferma restando la condizione di cui sopra), ove una di tali proposte fosse approvata, il parere è da intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle restanti».

ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.0.200, 3.0.201, 3.0.202, 3.0.203 4.0.200 sono improponibili, perché estranei al contenuto del disegno di legge in esame, recante disposizioni in materia di «Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo».

il mio Gruppo sta dando indicazione di astenersi dal voto, vorrei precisare che, in maniera non conforme al Gruppo a cui appartengo, voterò a favore dell'articolo

a quello che propone una norma valida per tutti gli istituti culturali, che non ne privilegi alcuni e ne lasci morire altri, come invece accade con questa norma, che pure riguarda istituti di cui - ripeto - apprezziamo l'attività. Voglio ricordare al Governo che in Commissione non abbiamo ancora potuto discutere

si introducessero criteri trasparenti, validi per tutte le istituzioni culturali. L'Accademia della Crusca, come già detto, è una delle istituzioni più importanti sullo studio, la storia, la promozione e la diffusione della nostra lingua.

emendamenti. Spiace che la Presidenza li abbia ritenuti estranei alla materia, perché queste istituzioni fanno anche studi sulla parte medievale di loro competenza. Quindi, ci sembra un po' forzata l'interpretazione della Presidenza; comunque, questa è, e noi la accettiamo per quella che è, pur non condividendola. Mi auguro che almeno il Governo voglia tenere conto dei contenuti dei nostri emendamenti, che non sono pretestuosi ma sono davvero a favore delle istituzioni culturali di eccellenza del nostro Paese. finestra") *(PD)*. Signora Presidente, anch'io mi dissocio dall'interpretazione data dalla Presidenza su questo provvedimento, perché di istituzioni culturali stiamo parlando e gli emendamenti erano inerenti alla materia. Il mio emendamento, il 3.0.201, in particolare riguarda la richiesta di un contributo a favore dell'Accademia dei Lincei.

della Crusca e su quella dei Lincei, ovvero su un concetto più generale, quello di ampliare il contributo a tutte le istituzioni culturali per poi delegare al Governo un'oggettiva ripartizione si erano create le condizioni per andare avanti. Il Governo evidentemente non ritiene l'Accademia dei Lincei e neanche quella

queste importanti istituzioni culturali. Ha fatto una scelta di chiusura, dal nostro punto di vista incomprensibile, però, contemporaneamente, il Ministro

grazie all'attenzione che il Presidente riserva proprio all'Accademia dei Lincei e all'Accademia della Crusca). Non comprendiamo l'atteggiamento del Governo, e neanche quello di questa maggioranza, che ha voluto perseverare nell'escludere

aggiungere degli "spiccioli" e sanare delle situazioni molto complesse, in questo 2011, che è un anno molto particolare. Continuiamo a criticare fortemente il Governo per questa assenza e latitanza, per questa mancanza di sensibilità,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, in questa mia breve dichiarazione di voto non posso che confermare il giudizio positivo espresso già in discussione generale su questo disegno di legge.

mondo, per definire la nostra identità e il nostro ruolo nel mondo. Pensate ad esempio che negli Stati Uniti d'America il numero di studenti che frequentano gli istituti di lingua italiana sta aumentando in modo vertiginoso e ciò significa diffondere la nostra identità e i nostri valori anche nel Nord America. Pensate, per esempio, che la Cina sta trasformando il suo diritto privato ricorrendo a studiosi italiani di diritto romano. Ciò significa ancora una volta che le politiche culturali possono svolgere un ruolo fondamentale anche nella politica estera. Con riferimento poi al finanziamento della cultura

ma è proprio in tale contesto che dobbiamo fare ciò che è stato fatto da tempo in altri Paesi e cioè coinvolgere i privati con adeguate politiche fiscali che li incoraggino a intervenire e a sostenere la cultura anche in Italia. Ovviamente, laddove si tratti di istituzioni e di fenomeni culturali di particolare significato per l'identità, la storia e lo sviluppo del nostro Paese, lo Stato non può cessare di fare la propria parte.

che porti a evitare scelte politiche nella individuazione degli istituti culturali da finanziare, come troppo spesso maggioranze di colore diverso hanno fatto sia di sinistra, che di centro e di destra. Non dobbiamo finanziare gli enti e gli istituti amici, ma chi svolge un ruolo importante, chi fa qualità di ricerca e diffusione di sapere. selezione degli interventi e meritocrazia anche in questo settore, alla luce di un'importante e significativa riforma della legge 534. Mi associo poi anch'io, proprio nella ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia,

l'attenzione alla nostra lingua italiana, proprio in un momento in cui, fra l'altro, l'eredità linguistica è cemento sempre più forte di un'unità nazionale che è fondamentale per poter consentire al nostro Paese di recuperare quell'orgoglio che gli consenta di affrontare momenti difficili che soltanto con una forte coesione e una forte consapevolezza del nostro essere italiani, della nostra storia e della nostra identità possiamo superare.

auspicando che non sia soltanto un'occasione isolata e che sui grandi temi che dividono spesso questo nostro Paese ci possa essere, torno a ribadire, una concordia che presuppone una maggiore disponibilità e sensibilità del Governo a ascoltare il Parlamento e a venire incontro ad esigenze ampiamente

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, illustri colleghi, approda in Aula il provvedimento con cui si procede all'erogazione di contributi agli enti di ricerca sul Medioevo. Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare consta di sei articoli, quattro dei quali relativi al finanziamento di altrettanti enti di ricerca.

ha esaminato spesso con grande attenzione il tema relativo alle politiche culturali; come diceva la senatrice Vittoria Franco poc'anzi, avevamo approvato anche un ordine del giorno all'unanimità. Troppo spesso però i provvedimenti che

l'Istituto storico italiano per il medio evo, il Centro italiano di studi sull'alto medioevo, nonché l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia. I due articoli rimanenti concernono la copertura finanziaria e le disposizioni finali. Con riferimento alla prima, ovvero alla copertura finanziaria, di cui all'articolo 5, l'onere è quantificato in 2.070.000 euro a decorrere dal 2012, che si prevede di coprire mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,

che meritano adeguata attenzione e adeguato rispetto. Non si può procedere prescindendo da un contesto globale, senza quindi analizzare l'insieme con la giusta attenzione e con il giusto rispetto. Ma questo - purtroppo, ci stiamo abituando - è l'atteggiamento dominante

a nostro avviso l'assoluta inadeguatezza culturale e politica di questo Governo. Riconosciamo come certamente importante il ruolo di questi quattro istituti. Lo abbiamo detto e lo continuiamo a sostenere in quest'Aula: si tratta di quattro istituti importanti, che svolgono un lavoro importante, a cui va il nostro riconoscimento. Andava fatta però una ricognizione delle eccellenze, che rappresentano per il nostro Paese dei patrimoni imprescindibili: ce ne sono tante che oggi rischiano di essere mortificate e non valorizzate. legge n. 2548 si dispongono contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del Medioevo italiano ed europeo, attribuendo risorse per sostenere istituti che svolgono attività attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura latina del medioevo, elevandoli fortunatamente al rango di utili mezzi culturali per il nostro Paese. Perché sceglierne solo quattro e mortificarne tanti altri? Questi istituti rappresentano un importante patrimonio: lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Sarebbe stato sicuramente meglio prevedere che detti contributi fossero erogati dall'Esecutivo con atti differenti dalla legge, e che, per individuare tutti gli enti da enti da finanziare, fossero stabiliti determinati requisiti ai fini dell'accesso al contributo. Avremmo preferito di gran lunga un disegno di legge più snello, contenente i criteri da rispettare e i requisiti da soddisfare al fine di avere accesso ai contributi suddetti per tanti e diversi enti che espletano ricerca sul Medioevo, contributi che avrebbero potuto meglio e di gran lunga superare le briciole concesse "ad entem" È apprezzabile l'iniziativa (l'abbiamo detto e lo confermiamo in questa sede), ma non la *ratio* di base, che porta all'individuazione soltanto di qualche istituto. Anche in questa occasione avete perso un'importante occasione.

per voi le politiche culturali e le politiche legate al mondo della scuola, dell'università e della ricerca sono marginali rispetto alle politiche economiche e di bilancio. Noi a tutto questo non ci stiamo, e vi confermiamo oggi il nostro voto di astensione su un provvedimento che non condividiamo nel metodo, ma che condividiamo nel merito. L'astensione dell'Italia dei Valori non è certamente diretta ad ostacolare i finanziamenti: essa è invece da ricondurre alle modalità di attribuzione degli stessi, a quella selezione naturale che con il presente disegno di legge viene posta in essere includendo o escludendo questo o quest'altro degli istituti ai fini

signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, abbiamo votato a favore di tutti gli articoli di questo provvedimento e voteremo ovviamente anche a favore del disegno di legge Condivido le perplessità alle quali il relatore ha fatto riferimento,

riconoscimento. È vero che qualcuno potrà contestare il fatto che altre istituzioni restano fuori da questa contribuzione. Quante volte, però, si è invocato il tema della scelta e delle priorità come elemento che qualifica la politica? Questo è, e questo mi pare che in questa giornata venga fatto. Certo, ci dispiace che non sia stato fatto uno sforzo suppletivo.

lingua italiana, quella ordinata dall'«uomo di Firenze», come dice una bella canzone, potesse avere un riconoscimento per il grande lavoro che in questo momento viene fatto dal Centro Pio Rajna per costituire una bibliografia di prima grandezza. Si tratta d'altra parte di rivolgere attenzione a quel patrimonio così fondamentale e formidabile qual è il patrimonio immateriale di cui la nostra cultura si può avvalere.

lo studio del Medioevo consenta di conoscere bene la nostra civiltà, come ogni buono studio del passato permette di conoscere bene il presente

fra molti numeri e molti conti che sembrano non tornare mai, l'aver privilegiato l'attenzione ed il contributo per le parole, per le nostre parole - che forse ci aiutano

il provvedimento sul quale ci accingiamo a votare è volto a sostenere quattro istituti di ricerca di importanza internazionale nel settore degli studi medievali. La 7a Commissione ha ha effettuato un attento esame delle loro caratteristiche, della specificità che distingue ognuno di essi, della vastità della loro produzione scientifica e delle esigenze che ne conseguono per assegnare i contributi destinati a fornire una base stabile per articolare progetti di ricerca in un orizzonte temporale adeguato. Il provvedimento è stato elaborato con una visione complessiva dell'intero settore di studi interessato all'intervento, in una prospettiva che rispetta l'autonomia degli istituti, ma prefigura uno scambio di informazioni e una cooperazione scientifica che potrà razionalizzare l'impiego delle risorse e accrescere la qualità e il valore dei risultati in esse contenuti. Si è richiesta anche, mediante annuali rendiconti, un'assunzione di responsabilità rispetto all'impiego dei contributi concessi, per assicurare la loro effettiva destinazione alle attività istituzionali e l'efficacia del loro impiego. Una visione parziale del Medioevo l'ha definito come l'epoca della decadenza e delle barbarie. La ricerca su storia e cultura del Medioevo italiano ed europeo ha dimostrato al contrario l'importanza di inserirci nel solco della nostra storia, per recuperare la nostra identità: operazione fondamentale per mettere correttamente a fuoco il nostro presente. La Lega Nord intende fornire il proprio contributo per consentire agli istituti che studiano il Medioevo di superare problemi finanziari, organizzativi e strutturali. Dichiariamo quindi il voto favorevole al provvedimento.

la cultura non entra nelle discussioni dell'Aula all'interno di provvedimenti o manovre economiche che prevedono tagli di risorse, scioglimenti di enti di grande rilevanza. D'altra parte, però, già nell'intervento del relatore e in quelli in Commissione suscita evidente perplessità la scelta di ricorrere ad uno strumento normativo primario, come il disegno di legge, per restituire risorse precedentemente ridotte a quattro enti che svolgono ricerche sul Medioevo, quali la Società internazionale per lo studio del medioevo latino (600.000 euro), la Fondazione Ezio Franceschini (450.000 euro), l'Istituto storico italiano per il medio evo (500.000 euro), nonché il Centro italiano di studi sull'alto medioevo (450.000 euro), contributi che peraltro gli enti suddetti potranno ricevere solo a partire dal 2012. Si tratta di enti la cui attività è particolarmente importante per quanto il Medioevo rappresenta nella storia della cultura, dell'arte e religiosa del nostro Paese, dunque non vi è dubbio che da parte del nostro Gruppo si ritenga opportuno il ripristino di queste risorse. Ma perché non inserire questi contributi all'interno di una riflessione generale sugli istituti culturali che beneficiano della legge n. 534 del 1996? Perché non prendere nemmeno in esame i nostri emendamenti che chiedevano di includere le Accademie della Crusca e dei Lincei tra i beneficiari di questo provvedimento? Parliamo in questo caso di enti che diffondono la cultura e la lingua italiana in tutto il mondo. Perché non ragionare dunque su un progetto? Perché questa idea di selezionare arbitrariamente enti meritevoli da altri altrettanto meritevoli, se non per scegliere, secondo l'espressione - infelicemente attribuita a Giolitti - per cui le leggi con gli amici si interpretano, con gli altri si applicano. Siamo dunque costretti a distinguerci con un voto di astensione, perché nel merito c'è la nostra soddisfazione per il reintegro delle risorse per enti di importante rilevanza storica e culturale, nel metodo vi è l'uso di uno strumento improprio. Non deve infatti sfuggire all'attenzione di tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, che nelle stesse condizioni in cui si trovano questi quattro enti si trovano attualmente moltissimi altri istituti nazionali che, pur di fronte ad una meritoria e apprezzata attività culturale che qualifica anche all'estero la civiltà del nostro Paese, si vedono decurtato il contributo statale per il 2011 per una percentuale che oscilla tra il 20 e il 50 In conclusione, si auspica che, a partire dal libro bianco a cura dell'Istituto storico italiano per il medio evo, dal significativo titolo - lo ricordo al Governo - "Medioevo negato", il Governo e la maggioranza prendano finalmente consapevolezza che la cultura è un investimento fondamentale per questo Paese e merita quell'attenzione e quelle risorse

ringrazio il relatore e il Governo per i loro interventi e per l'attenzione che questo provvedimento, anche se di natura parlamentare, pone a livello culturale, anche se in un settore specifico, quello dell'Alto medioevo. qualcuno ha ricordato precedentemente i contributi ai quattro enti, ma ha dimenticato, a mio parere, una cosa importante, il quinto contributo, pari a 70.000 euro, che riguarda l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (cioè, si pone mano alla conservazione e pubblicazione dei testi latini che vanno dal V al XV secolo,

particolarmente significativo che questa attenzione sia rimasta inalterata. Vorrei dire, in conclusione, che è fuori di dubbio che questo provvedimento abbia destato alcune perplessità, perché avremmo preferito che fosse il Governo stesso ad intervenire, per quello che era possibile,

boicottare questo provvedimento, non vararlo, significava infliggere anche a questi enti sull'Alto Medioevo la morte certa. Oggi finalmente avranno un finanziamento sicuro e costante nel tempo, che è fondamentale per questi istituti, per poter programmare la loro attività futura. È un pozzo di storia culturale del Paese, fondamentale per l'Italia, per l'Europa, ma anche per il mondo intero. per il mondo intero. È indubbiamente vero che avere queste fondazioni, questi enti di ricerca, questi enti di cultura può portare,

che il consenso fosse stato anche qui ben più ampio. Apprezzo l'astensione di alcuni colleghi dell'opposizione; apprezzo di più chi voterà favorevolmente.

in dissenso dal Gruppo, il mio voto favorevole. Condivido pienamente l'analisi che il Gruppo del Partito Democratico ha fatto sulla materia. È chiaro che qui urge una normativa di carattere generale che ricomprenda tutti gli enti, segnatamente alcuni enti dell'importanza dell'Accademia della Crusca. Tuttavia ritengo che questi soggetti a cui oggi si riferisce il disegno di legge abbiano una dimensione non solo nazionale, ma addirittura internazionale. Proprio in questi giorni in cui le controversie tra noi e la Germania sono sotto gli occhi di tutti, mi premerebbe dire una cosa: se la Germania avesse solo uno di questi enti, sicuramente non starebbe a disquisire su quali e quanti contributi debbano essere assegnati. Permettetemi poi, poiché il senatore Benedetti Valentini ha ricordato un insigne medievista, di ricordare qui un altro medievista, il professor Ezio Franceschini, di cui mi onoro di essere stata allieva, che ha reso grande la storia della letteratura medioevale latina nel nostro Paese. A lui è intitolata una fondazione che promuove, soprattutto, lo studio di queste materie, attraverso un numero grandissimo di giovani.

Per tutti questi motivi, non posso che ribadire il mio voto favorevole a questo provvedimento, dichiarando, tuttavia, che non è possibile che in un Paese come il nostro, proprio sulle istituzioni di grande cultura si debba ogni volta distinguere tra una e l'altra senza mai entrare nel merito e senza mai chiederci veramente e fino in fondo quali sono gli istituti che rendono grande il nostro Paese, non solo qui, tra gli studiosi italiani, ma soprattutto all'estero. Mi auguro pertanto che a questo provvedimento ne seguano altri che ricomprendano gli istituti qui citati

desidero informare l'Aula che voterò in dissenso dal mio Gruppo, ma non vorrei essere frainteso. Infatti, condivido

conoscere la nostra storia, le nostre radici. Purtuttavia, non riesco a comprendere, innanzitutto, che cosa ancora ci sia da ricercare sul Medioevo. Per dirla francamente, vi sono centinaia di migliaia di studi, pubblicazioni e libri che da trecento da trecento anni riempiono le biblioteche e che godono di una discreta consultazione. L'importanza di conoscere la propria storia si esplica nello studiare la storia, non continuando per centinaia di anni a fare ricerca. In secondo luogo, l'Italia dedica certamente poche risorse alla ricerca,

per sostenere quattro istituti che fanno ricerca su tale periodo, ricerca che, tra l'altro, viene svolta anche da tanti altri enti a livello universitario.

se c'è un periodo durante il quale la nostra storia ha ben poco prestigio è proprio il Medioevo. Quindi, potremmo anche concentrarci a diffondere i grandi valori della nostra cultura là dove sono veramente grandi. grandi. Ribadisco che considero estremamente importante la cultura, ma non condivido questo disegno di legge. Quindi,

Il Senato, premesso che: la promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo ha subito con i provvedimenti di natura finanziaria adottati dal Governo dal 2008 ad oggi tagli in particolare, l'Accademia nazionale della Crusca svolge un ruolo prezioso in Italia e nel mondo quale punto di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana; l'Accademia nazionale della Crusca sostiene l'attività scientifica e la formazione di nuovi ricercatori nel campo della linguistica e della filologia italiana, acquisisce e diffonde, nella società italiana e in particolare nella scuola, la conoscenza storica della nostra lingua e la coscienza critica della sua evoluzione attuale, collabora con le principali istituzioni affini di Paesi esteri e con le istituzioni governative italiane e dell'Unione europea per la politica a favore del plurilinguismo del nostro continente; anche l'Accademia nazionale della Crusca, come molti altri istituti culturali del nostro Paese, ha visto ridurre in questi ultimi anni, le risorse necessarie a garantire il suo funzionamento e la sua stessa sopravvivenza, impegna il Governo a reperire le risorse per garantire ad un'antichissima istituzione la possibilità di continuare a svolgere il suo importante ruolo in Italia e nel mondo.

il tema che oggi affrontiamo ha avuto una lunghissima gestazione: quasi 20 anni di dibattito, di leggi importanti, ma mai attuate definitivamente. Stiamo parlando del riordino delle professioni sanitarie, nello specifico dell'istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Parliamo complessivamente di 22 nuove professioni sanitarie e di oltre 500.000 operatori, per i quali l'*iter* del percorso di organizzazione delle professioni è iniziato con la legge n. 502 del 1992, proseguendo con la legge n. 251 del 2000 fino alla legge n. 43 del 2006. Quest'ultima ebbe il grande merito...

e, attraverso una delega al Governo, di istituire appositi ordini professionali in campo sanitario. Queste importanti innovazioni non hanno mai visto la luce e le deleghe al Governo, nei diversi passaggi della XIV legislatura, sono di fatto scadute.

Provvedimenti non adeguati avevano nel tempo creato disparità, commistioni tra dispositivi di principio e norme di dettaglio, l'assenza di un filo condutture legislativo moderno e al passo con i tempi e con le sempre maggiori richieste di sviluppo provenienti dal cittadino utente. Era arrivato il momento di eliminare le disparità di trattamento tra le diverse professioni sanitarie già organizzate in ordini e collegi, capaci per proprio ordinamento e finalità di fare una priorità della lotta all'abusivismo, una piaga una piaga purtroppo ancora molto presente, e nel contempo realizzare una vera promozione della qualità delle prestazioni sanitarie erogate. Con il disegno di legge in esame, agli ordini già riconosciuti si aggiungono cinque nuovi profili sanitari. Si riconoscono gli stessi compiti di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e di garanzia della qualità delle prestazioni nei confronti del cittadino. Si conferma la natura giuridica degli ordini quali enti pubblici non economici, a carattere nazionale, ausiliari dello Stato, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e organizzativa, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Il testo che andiamo ad approvare è formato da 19 articoli. Signor Presidente, ne dettaglierò soltanto alcuni, rimandando al successivo dibattito l'approfondimento degli altri. Il primo istituisce i cinque ordini: infermieri professionali, ostetriche, professioni sanitarie della riabilitazione, tecnici sanitari di radiologia medica, professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione. L'articolo 2 istituisce la consulta regionale degli ordini provinciali; l'articolo 3 istituisce per ogni ordine gli albi professionali; l'articolo 5 prevede la commissione disciplinare; l'articolo 8 prevede i requisiti per l'iscrizione all'albo.

Signor Presidente, il voto unanime della Commissione sanità del Senato - e mi auguro che così sarà anche in questa Aula - segna un passo importante, una risposta efficace, in tempi così difficili della politica, alle istanze dei professionisti sanitari e del cittadino utente, sempre più, giustamente, esigente.

Ringrazio il presidente Tomassini, che si è sempre battuto per ovviare a queste carenze, la senatrice Bassoli e tutte le opposizioni che, dentro una discussione ampia e franca, hanno permesso il varo di questo disegno di legge in Commissione sanità con voto unanime. Ora il passaggio in Aula consegnerà al Ministro la grande opportunità di porre la parola fine a una problematica rimasta aperta per troppi anni.

con la società civile, che in modo instancabile ha seguito questo provvedimento e ci ha accompagnato ed aiutato anche a migliorarlo nelle diverse espressioni delle professioni che sono qui riconosciute.

le sue radici legislative sono antiche, questo provvedimento trova però le sue ragioni vere non in un una abitudine parlamentare di accondiscendere a quanto succede nella società (cosa pur non scandalosa nel momento in cui si sviluppa un confronto corretto), ma affonda le sue ragioni nella trasformazione profonda che, nell'ambito medico e anche nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, hanno avuto queste professioni. La professione infermieristica, per esempio, si è evoluta tantissimo nel corso degli anni

si è passati dal diploma alle lauree brevi, e quindi si tratta, a tutti gli effetti, di laureati. Inoltre, la loro professionalità è cresciuta: è cresciuta: ad esempio, per quanto riguarda le professioni infermieristiche, tanti compiti che alcuni anni fa erano svolti dai medici oggi sono svolti, con grande professionalità, dagli infermieri professionali. Questo è un dato di cui, secondo me, dobbiamo tenere conto. C'è poi anche un'altra ragione che accompagna questo provvedimento, non solo la maggiore professionalizzazione e la maggiore formazione che queste figure hanno subito: vi è anche l'aspetto di tipo Sono figure che fino a poco tempo fa erano prevalentemente legate all'attività dipendente ospedaliera; oggi, invece, si tratta di figure (anche quelle infermieristiche ed ostetriche, ma soprattutto quelle tecniche) che hanno un'intensa attività libero professionale, e non solo come lavoratori dipendenti, sappiamo che gli ordini sono nati in prima istanza proprio per ordinare e garantire figure che si muovevano nell'ambito libero-professionale del nostro Paese.

dentro un ordine, passando dall'organizzazione spontanea dei collegi - perché queste figure professionali oggi sono ordinate dentro collegi, cioè ambiti privatistici e volontari

L'ordine, da questo punto di vista, garantisce una maggiore trasparenza e una migliore garanzia anche per il cittadino, sia per colui che viene assistito nell'ambito di un ospedale pubblico o privato accreditato, sia per chi deve scegliere il professionista sul libero mercato.

in generale, vorrei che la società non fosse complessivamente sottoposta a rigide regole di mercato: dobbiamo riscoprire anche gli aspetti umani, relazionali, professionali e formativi. C'è una ricchezza della società che va messa in evidenza, e la politica deve aiutare queste professionalità e gli elementi vivaci della nostra vita sociale ad emergere,

le corporazioni erano tipiche della società medioevale, erano organizzazioni privatistiche. Chi era più forte riusciva ad ottenere di più, chi era più debole otteneva di meno: anche dentro le corporazioni le logiche erano quelle della forza. Il passaggio dalla logica un po' più corporativistica quale quella del collegio, alla logica ordinamentale e pubblica sta anche in questa ricchezza, cioè nella capacità di garantire maggiormente la presenza e la forza nella contrattazione di queste professioni

ritengo che il disegno di legge che ci apprestiamo a votare sia un arricchimento per il nostro Sistema sanitario nazionale, dia una maggiore sicurezza per le cure e assicuri un maggiore riconoscimento della professionalità di alcune figure che nel corso degli anni hanno arricchito il loro percorso professionale.

fermiamoci di fronte all'atto che stiamo per fare al Senato della Repubblica. Fra l'altro, con un'incredibile e paradossale coincidenza di tempi rispetto a ciò che abbiamo esaminato con la manovra economica la settimana scorsa al Senato e che

gli ordini professionali non sono la soluzione rispetto alla possibilità di accesso al mercato, di garanzia dell'utente e dei consumatori, e contemporaneamente al Senato decidiamo di istituire ben cinque nuovi ordini professionali, nella materia delle professioni sanitarie, e ben 20 albi professionali che, in base all'articolo 11, in automatico potranno diventare 20 nuovi ordini.

dell'Aula. Poco fa il senatore Bosone parlava del riconoscimento di queste figure professionali, riconoscimento che anche noi vorremmo dare agli infermieri, alle ostetriche, al podologo,

delle corporazioni. Credo che nel 2011 forse si possa passare attraverso altre modalità. L'ordine garantisce innanzitutto la sua esistenza e l'iscritto all'ordine. La formazione ed anche il libero accesso alla professione, invece, sono a tutela ed a garanzia dell'utente, di chi appunto si troverà ad avere a che fare con questi professionisti. Le liberalizzazioni, che appunto si elogiano nei decreti a Ferragosto e che poi si smentiscono nelle Aule parlamentari il giorno dopo, non devono avvenire sempre a casa di qualcun altro: sembra che qui siamo tutti per le liberalizzazioni, le si attuano nel mercato dei taxi, i tassisti si ribellano; se si fanno per le farmacie, i farmacisti scendono in piazza; se si fanno per esempio per gli avvocati, gli avvocati, questi ci hanno mostrato con la riforma della professione forense che cosa sono in grado di fare: una riforma della professione forense che abbiamo esaminato in quest'Aula parlamentare che addirittura fa dei passi indietro rispetto alla legge fascista che aveva istituito l'ordine forense. Le liberalizzazioni, Le liberalizzazioni, per esempio, passano da queste Aule parlamentari per intervenire nel campo dell'editoria, e incredibilmente fanno l'operazione opposta, e quindi, per cercare di favorire il mercato

a fermarsi su questo disegno di legge. È davvero paradossale che in questo momento di difficoltà economica, mentre si si parla di fare riforme strutturali, addirittura costituzionali per cercare di rivedere l'impianto della nostra economia e ridare slancio al Paese, un Paese che tutti riconosciamo essere frenato e bloccato dai vincoli e, sì, proprio dalle corporazioni, al Senato decidiamo di istituire cinque nuovi ordini e venti albi che potrebbero diventare altrettanti ordini professionali. un sussulto di dignità potrebbe far sì che l'Assemblea si fermi un attimo. Spesso viene sostenuto che l'ordine professionale serve all'utente, al consumatore e al cittadino per avere dei professionisti

«un percorso formativo di livello universitario obbligatorio, come peraltro ribadito in materia dalla Commissione europea, da ultimo nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del febbraio 2004».

Quando un'Autorità sottolinea queste cose e chiede al legislatore, in una nuova indagine sugli ordini professionali del 2009, di evitare l'istituzione di nuovi ordini professionali

altrimenti potremmo anche decidere di abolirla. Ogni volta che citiamo i pareri e le indagini che porta avanti l'Autorità *antitrust*, infatti, il Governo e il Parlamento sembrano assolutamente essere sordi ai suoi richiami.

Il mercato può avere le sue regole e cercare di favorire tutti quelli che sono presenti e che in qualche modo vedono

logopedisti, fisioterapisti, podologi, infermieri, dietisti e igienisti dentali,

suggerirei quanto meno di rileggere la manovra economica che hanno licenziato la settimana scorsa al Senato e che in queste ore è all'esame della Camera dei deputati. Lì enunciate il principio delle liberalizzazioni, sottolineate che gli ordini professionali possono essere qualcosa di negativo per l'accesso al mercato, che gli ordini devono aprirsi, enunciate tanti bei principi ma poi, un attimo dopo, andate esattamente nella direzione opposta. Per quanto ci riguarda abbiamo presentato come Radicali degli emendamenti, anche se il testo è "inemendabile", e infatti i nostri emendamenti sono semplicemente e meramente di tipo soppressivo. Abbiamo anche presentato un ordine del giorno con in cui vi richiamiamo non soltanto il parere dell'*Antitrust*, ma anche il testo testo della manovra in discussione in queste ore. L'appello che vi faccio in questo momento è davvero di fermarvi un attimo e di ripensare se davvero l'ordine professionale nel 2011 sia l'unica garanzia per l'utente e il consumatore, anche nel settore della sanità.

la questione della regolamentazione e del riordino delle professioni sanitarie approda nell'Aula del Senato. Al contrario di quello che può essere l'atteggiamento di alcuni organi di stampa, avversi a questo provvedimento, noi dell'Italia dei Valori riteniamo che l'obiettivo di questo disegno di legge sia volto prioritariamente a tutelare l'interesse del paziente e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate e non interessi di tipo corporativistico dei professionisti. Piuttosto che un ordine di tipo tradizionale, ritengo che questo provvedimento tenda ad istituire un vero e proprio pubblico registro degli operatori delle varie professioni sanitarie. È il primo e importante passo verso la conclusione positiva di una vicenda dipanatasi in maniera alquanto complessa e travagliata attraverso tre legislature.

tecnico-sanitarie e della prevenzione i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione. Purtroppo, come molti colleghi sanno e come sicuramente sanno i tanti operatori delle professioni sanitarie, alla legge n. 43 del 2006 non è mai seguita la decretazione legislativa prevista della delega contenuta all'articolo 4 della legge stessa. Nonostante la allora concorde volontà degli schieramenti di maggioranza ed opposizione, nella scorsa legislatura non solo non si è provveduto a disciplinare il settore, ma si è anche lasciata decadere la delega prevista nell'intervento legislativo tutt'ora in vigore. Già sul nascere di questa legislatura sorgeva, quindi, la necessità di prevedere un disegno di legge ordinario che definisse esaurientemente le professioni sanitarie, la loro distribuzione in ordini professionali e la corretta collocazione in questi ultimi degli albi professionali, prevedendo altresì la dislocazione territoriale degli ordini, gli organi di questi ultimi, le loro attribuzioni, le modalità di elezione, i rapporti tra gli ordini e la pubblica amministrazione, la disciplina degli albi professionali, i requisiti per l'iscrizione al loro interno e le federazioni nazionali degli ordini, con relativi organi A tal fine, avevo presentato a mia firma un disegno di legge (che è stato poi fatto proprio dal mio Gruppo) con il quale si intendeva dare una compiuta ed organica regolamentazione alla materia. Non posso tacere qui un certo rammarico per il fatto che questo disegno di legge sia stato rapidamente accantonato da parte della Commissione sanità. Se è pur vero che molte delle indicazioni in esso contenute sono state di fatto poi recepite attraverso vari ordini del giorno, continuo a ritenere che quel quel disegno di legge avrebbe potuto dimostrarsi maggiormente soddisfacente e definire in maniera più completa ed organica l'intera materia. In esso infatti si prevedeva l'istituzione di sette ordini, ivi compresa la trasformazione dei collegi già esistenti, ossia infermiere, ostetrica e tecnico di radiologia. Il testo del quale discutiamo oggi in Aula è comunque un buon risultato; è necessario ora il massimo impegno di tutte le forze parlamentari affinché l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento porti ad una rapida approvazione definitiva, soddisfacendo così le attese di circa 600.000 professionisti L'esigenza prioritaria, del resto, rimane quella di assicurare la soddisfazione del paziente. Ciò è possibile anzitutto favorendo il superamento della disparità di trattamento tra le professioni sanitarie già organizzate in ordini e collegi e quelle che ancora non presentano tale articolazione. Tale intervento è infatti destinato ad influire positivamente sia sulla lotta all'abusivismo, che nel settore in esame continua ad essere elevatissimo, sia sulla promozione della qualità delle prestazioni erogate e del massimo livello di professionalità. Questo disegno di legge costituisce un primo passo per la soddisfazione delle giuste esigenze di tutte le categorie, le quali potranno finalmente trovare una loro propria e definitiva regolamentazione. A tal proposito, voglio ribadire nuovamente la necessità, da me già sostenuta nel corso del dibattito in Commissione, di un riposizionamento della figura del tecnico ortopedico nelle professioni sanitarie dell'area riabilitativa. Il profilo professionale del tecnico ortopedico, infatti, ha consolidato il suo ruolo nel panorama sanitario, identificandolo quale parte attiva del trattamento multidisciplinare previsto nel piano riabilitativo del paziente. ministeriale n. 665 del 14 settembre 1994, il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o l'adattamento, l'applicazione e la fornitura di protesi, di ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore. L'attuale inserimento del tecnico ortopedico nella classe delle lauree in «professioni sanitarie tecniche» non riflette quindi, a mio avviso, il ruolo svolto dai suddetti operatori all'interno del sistema sanitario, ruolo di estrazione puramente riabilitativa. Sfido chiunque, infatti, a riabilitare un paziente affetto da patologie o traumi dell'apparato locomotore senza l'opera insostituibile del tecnico ortopedico. Insieme ad altri colleghi ho a tal proposito sottoscritto uno specifico ordine del giorno (che il Governo ha accolto in Commissione), volto a favorire il riconoscimento della professione del tecnico ortopedico come professione sanitaria dell'area riabilitativa. Concludo, colleghi, affermando che sicuramente avremmo potuto fare di più e in tempi molto più brevi. Mi auguro ora che l'altro ramo del Parlamento colga l'urgenza che sottintende questo provvedimento e proceda ad una rapida approvazione, per dare quantomeno eguale dignità lavorativa alle diverse professioni sanitarie e soprattutto garantire all'utenza la massima professionalità.

il provvedimento in esame assume particolare rilievo in quanto la creazione di ordini professionali in campo sanitario è positiva non solo per il riconoscimento di specifiche professionalità, ma anche come strumento di maggiore tutela e garanzia per il cittadino paziente, soprattutto quando questi vi ricorre direttamente in ambito di libera professione. Va sottolineato inoltre che questo provvedimento è stato molto discusso in Commissione sanità. Cito ad esempio, a riprova di quanto detto, la proposta emendativa formulata dall'opposizione e finalizzata ad una modernizzazione degli ordini attraverso uno scambio di informazioni sia tra sia tra i professionisti stessi, sia tra costoro e l'utenza destinataria delle loro prestazioni. Io spero che si comprenda lo spirito costruttivo di questo disegno di legge. Certamente nel corso di questa discussione in Aula potranno emergere ulteriori proposte migliorative, ad esempio per quanto riguarda l'attività di aggiornamento e formazione professionale dei propri iscritti; il ruolo che deve essere riconosciuto agli ordini va incrementato, sottolineandone il ruolo centrale. Su questo tema lo stesso Presidente della Commissione ha auspicato un'ampia ed approfondita riflessione in Assemblea. Tutto si può migliorare. Un ulteriore elemento di positività è costituito a mio giudizio dal fatto che con la creazione degli ordini professionali viene offerta una garanzia di maggior tutela del cittadino e, contestualmente, viene inferto un duro colpo all'abusivismo professionale: troppo spesso ci si imbatte in figure poco chiare che, facendo leva sullo stato di bisogno e di fragilità del paziente, ne approfittano in modo indebito a danno del paziente stesso, ma anche degli stessi ma anche degli stessi professionisti onesti, seri e preparati, facendo diminuire la fiducia delle persone nei confronti di intere categorie professionali. Infine, se sono vere - come lo sono - le mie considerazioni sin qui svolte, mi sia consentito esprimere anche un sentimento di amarezza: se è sicuramente positivo il riconoscimento ordinistico di queste professioni, gli ordini degli infermieri e di altre figure professionali

senatore Rizzi.

nella pienezza della loro competenza, andando quindi a creare un netto spartiacque tra i venditori di fumo, gli abusivi, che continuano a solcare il nostro territorio nazionale

delle due o tre professioni storiche del medico e dei cosiddetti paramedici. La scienza avanza, e questo disegno di legge, che speriamo diventerà quanto prima legge,

tutte le professioni sanitarie di cui si parla oggi e, in parziale contrasto con la senatrice Poretti, di cui ho ascoltato l'intervento in maniera molto interessata, preciso che non abbiamo fatto una legge per seguire gli interessi di qualcuno, ma abbiamo fatto una legge assieme a qualcuno: a coloro che hanno tutto il diritto di vedersi riconoscere la propria professionalità.

che però deve fare i conti con continui tagli alle risorse: basti pensare a cosa è accaduto nella penultima e nell'ultima manovra in materia di risorse in campo sanitario.

fra le Regioni del Nord e del Centro-Nord e quelle del Sud e del Centro-Sud, e viceversa. La popolazione invecchia, diminuiscono le malattie acute, aumentano quelle croniche, e quindi c'è bisogno di un personale sanitario preparato a far fronte a questo bisogno di continuità di cura. È necessario un personale addestrato ad utilizzare le nuove tecnologie, che cambiano quasi quotidianamente nel nostro sistema, un personale in grado di affrontare possibili gravi incidenti o crisi sanitarie pubbliche, come è avvenuto ultimamente rispetto all'H1N1.

un rischio clinico che ancora sottovalutiamo fortemente, ma che spesso è causa di situazioni molto gravi nelle nostre strutture sanitarie. Orbene, essendo questo lo scenario che abbiamo di fronte, dobbiamo valutare anche un altro elemento, ovvero il cambiamento del rapporto fra il paziente e le figure mediche e sanitarie. Non solo il paziente non vuole più essere definito tale, ma constatiamo anche che in questi anni è aumentato enormemente il contenzioso tra personale sanitario e pazienti, anche perché i progressi della medicina sembrano aver cancellato il concetto di morte Tutto questo comporta un costo economico

Per rispondere a queste sfide è necessario un personale preparato, efficiente ed efficace, che professionalmente sia all'altezza dei nuovi bisogni indotti dall'allungamento della vita, ma anche dalla crescente immigrazione e dalla necessità di cure continuative che danno a queste figure sanitarie un ruolo più ampio e qualificato. Infatti, anche se non sono figure mediche, e tradizionalmente vengono considerate ad un livello inferiore e comunque meno importante, oggi diventano importantissime nel processo di continuità di cura. la Commissione europea ha adottato nel 2007 il libro bianco dal titolo «Insieme per la salute» e nel 2008 un libro verde che mira a rafforzare la visibilità delle tematiche attinenti al personale sanitario e a verificare analogie tra le sfide che devono essere affrontate dal personale, i manager sanitari locali e quindi tutelare nella prospettiva la loro professionalità. Nel libro verde europeo si affronta il tema della formazione professionale permanente, poiché l'aggiornamento professionale contribuisce a migliorare la qualità dei risultati sanitari e garantire la sicurezza dei pazienti.

che, con le carenze di personale sanitario in molti Paesi europei, compresa l'Italia (ne parlava poco fa la senatrice Biondelli), diventerà sempre di più una tematica da considerare e da mettere in primo piano, insieme c'è il fatto che noi ormai ci apriamo a una libera circolazione dei pazienti, ma anche dei professionisti in questo campo. Ecco perché la discussione di questa normativa oggi dovrebbe darci l'occasione non tanto e non solo di dare una risposta inerente all'istituzione di ordini di alcune categorie sanitarie, ma anche per approfondire i temi inerenti alla costituzione di questi nuovi ordini, in grado quindi di rispondere a queste problematiche e a queste esigenze. Noi certamente avremmo voluto una legge più snella, e abbiamo cercato anche da questo punto di vista di dare un contributo nella Commissione. Avremmo voluto un numero minore di ordini, però la sintesi a cui siamo arrivati ci pare abbastanza soddisfacente. Certo, esprimiamo una preoccupazione: che, mentre si approva

usciamo da questa contraddizione tra il contenuto di una manovra, contro la quale peraltro abbiamo votato, e il testo che andiamo ad approvare in queste ore. Noi siamo per la liberalizzazione delle professioni: però, quando parliamo di professioni sanitarie, parliamo di attività che attengono ad un rapporto umano e professionale che deve essere improntato ad un'etica, ad una moralità e ad una professionalità che non devono essere comunque messe in discussione. Vorrei fare notare che questa esigenza non è solo nostra, perché in altri Paesi come la Francia esiste ad esempio un ordine degli infermieri e in Europa esiste un organismo federato della rappresentanza di alcune di alcune professioni sanitarie. Certo, veniva riportata dalla senatrice Poretti una frase del Garante della concorrenza e del mercato, che aveva espresso già un giudizio quando nel 2006 veniva data, attraverso una legge specifica, una delega all'allora ministro Turco per istituire questi ordini. Nel testo dell'ordine del giorno che è stato presentato dalla senatrice Poretti e altri e altri si dice che il Garante rilevava che la costituzione di nuovi ordini professionali e relativi albi potrebbe provocare una restrizione della concorrenza, a meno che - egli diceva, e questa mi sembra una questione importante su cui riflettere - non ci sia un'asimmetria informativa tra il consumatore e il professionista e sia necessario, al fine di garantire maggiori benefici al consumatore, consentire l'accesso a determinate attività solo a quanti possiedono specifici requisiti di qualificazione professionale. Ecco quindi che lo stesso Garante della concorrenza e del mercato ci mette che, se è vero che istituendo degli ordini si possono provocare anche delle restrizioni (e non è questo il caso), qualora si verifichi un'asimmetria informativa tra il consumatore - che io non vorrei fosse definito tale, perché noi non consideriamo la sanità un mercato

quelli esistenti. Quindi con queste valutazioni, credo sia anche importante pensare al fatto che non possiamo trasformare un sistema universale che garantisce a tutti il diritto alla salute, perché è un diritto

in questo caso, il rischio di danno per la salute delle persone più deboli è veramente molto grave. Naturalmente non parlo di chi sa difendersi perché ha gli strumenti economici e culturali

ma ritengo sia stato accolto un emendamento importante in Commissione che è un po' la chiave di come noi intendiamo oggi l'istituzione di questi ordini che adesso sono costituiti in collegi o albi professionali. Mi riferisco all'emendamento che obbliga gli ordini provinciali alla predisposizione di siti informatici attraverso i quali dare adeguata pubblicità alle proprie attività, alle attività formative, e che siano in grado di fornire l'elenco degli iscritti, compresi tutti i titoli con cui gli iscritti hanno diritto di accesso all'ordine, nonché le sanzioni disciplinari applicate agli iscritti nel caso in cui queste ci siano state nel corso della loro attività lavorativa. In sostanza, signor Presidente,

questa attività di formazione non può essere eseguita una volta per tutte: bisogna prevedere una formazione continuativa (noi abbiamo proposto almeno 50 ore annuali) di cui gli ordini si devono far carico, se vogliono essere ordini nuovi che non si istituiscono per salvaguardare un ordine corporativo, ma per dare esempio di professionalità, di qualità e per richiedere ai propri iscritti una professionalità e una trasparenza che tuteli l'interesse dei cittadini. Questi

Sulla liberalizzazione delle professioni già si è persa un'occasione, poiché la norma inserita nella manovra correttiva di luglio e poi ritirata dal Governo resta al palo. Vorrei richiamare l'essenza del problema. Una vera riforma delle professioni liberali si fonda sull'abolizione del valore legale del titolo di studio. Fino a quando non si porrà mano alla questione, ogni discorso sarà pura accademia. Infatti, come è evidente, non è il titolo di studio che ha intrinsecamente un valore legale, ma sono le conseguenze dettate da norme, regolamenti, organizzazioni che il possessore di esso è in condizione di fruire o sfruttare. Contro questo tipo di situazione si era schierata la norma proposta, appunto, nella manovra di luglio, che tagliava alla radice il bubbone corporativo degli ordini liberalizzando l'attività professionale. Il variegato fronte degli oppositori, in particolare la parte presente nelle Aule parlamentari, sostiene invece che, sì, le libere professioni intellettuali debbono essere riformate, ammodernando il sistema degli ordini ed eliminando le sacche corporative, tuttavia senza toccare il modello ordinistico, tant'è vero che nel provvedimento in esame si propongono cinque nuovi ordini e 20 albi. Io sono convinto, e lo dico da ingegnere di professione, che la legge così come era stata presentata a luglio era un'ottima scelta perché molto pratica, quanto è evidente che soprattutto in Italia, dove sullo stesso argomento ci sono molte posizioni diverse, ma, diciamo, almeno due opposte, è difficile immaginare una norma che salvi gli ordini e le sue prerogative e, al contempo, liberalizzi l'attività professionale. Dove si è tentata questa strada (ed è il caso dei servizi di ingegneria e architettura) esiste una confusione strisciante fra appartenenza agli ordini professionali e libertà di competere, con una mortificazione plateale delle norme ordinamentali, poiché le gare vengono assegnate, addirittura, su prezzi determinati (quelli di tariffa), ma con sconti anche dell'80 Mi auguro, pertanto, che si voglia ripensare questo provvedimento, che aumenta il numero degli ordini e degli albi e che dietro alla pretesa della tutela degli utenti aumenta questa società corporativa.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi senatori, naturalmente il tono assunto dall'ultimo spunto del senatore Menardi ci porterebbe a ragionare di altro: a parlare, probabilmente, come se il disegno di legge che

un mondo che non gradisce più essere considerato professionista di serie B. Non esiste la possibilità di immaginare percorsi di dirigenza alla pari nel momento in cui rimane l'assunto consolidato e scritto che alcuni sono professionisti veri, hanno un ordine e un albo e altri non lo sono. Quindi, il primo discorso - senatore Menardi, senatrice Poretti e colleghi

la relatrice questa sera ha sostenuto, che i proponenti del disegno di legge si sono proposti e che ha deliberato la Commissione igiene e sanità in modo ottimale, anche per il consenso che sta ottenendo in modo pressoché unanime da quest'Aula. Il primo passo è, pertanto, quello della pari dignità in un sistema che riteniamo costantemente di dover richiamare come sistema salute integrato. Un sistema dove la partecipazione delle forze, delle componenti, degli interessi, della ricchezza molteplice delle

Siamo abituati, ogni volta che si parla di accessi ai processi multidisciplinari, al letto del paziente, al capezzale dell'ammalato, ad immaginare solo medici. I mondi tecnico, professionale, infermieristico e delle altre variegate professioni che intorno alle necessità di salute si impegnano al letto dell'ammalato sono realmente diversificati e storicamente fondamentali e importanti. Nella realtà, sapete da quanto tempo abbiamo superato i mansionari? Oggi, se non facciamo questo, lasciamo i mansionari. La legge è cambiata. Il percorso è cambiato. Sono diventati professionisti, che hanno superato quel mansionario, che hanno un ruolo addirittura nella dirigenza, che le Regioni hanno fatto a gara a riconoscere, ma che deve essere ridato con la dignità propria anche dei titoli appropriati alle persone che, con studi diversi, abbiamo voluto che seguissero determinati percorsi e che da quelli professionalizzanti, che avevamo immaginato per tanto tempo, sono passati ai percorsi universitari, attraverso un processo organizzato dal Parlamento medesimo, che ha determinato la loro elevata professionalità. Oggi stiamo guadagnando al capezzale dell'ammalato non una scusante, caro senatore Menardi. Non stiamo dicendo che i pazienti sono un pretesto per una corporazione. Chi più di un medico vorrebbe sottolineare la differenza tra sè e chi c'è dopo? Ma sarebbe stupido e stolto da parte mia immaginare questo.

che tutti hanno rilevato frequentemente essere ricco di un abusivismo importante, che si presenta in diverse forme, da quello del terapista a quello dell'igienista dentale, a quello dell'infermiere. Oggi rimettiamo insieme questi dati, riconosciamo queste professionalità, le portiamo in un sistema di parità importante e concediamo che si possa naturalmente riconoscere questo lavoro che, per decenni, è stato promesso e che sta trovando una realizzazione in questo momento. Voglio cogliere anche l'occasione, vista la sensibilità del Ministro sull'argomento, è chiaro che tutto ciò non chiude, nell'ambito della disamina dei bisogni di salute, l'organizzazione sanitaria con cui dobbiamo affrontare Voglio ricordare che negli ultimi tempi si sta variegando una miriade di figure che talvolta sono riconosciute dalla Pubblica istruzione e non dal sistema sanitario; molte figure vengono riconosciute dall'una e non dall'altro. E nelle diverse Regioni, ora con una legge dell'uno e ora con una legge dell'altro, dell'altro, vengono integrate in un sistema di salute che, naturalmente, anche in quel caso non assicura una qualità controllata dal principio alla fine della loro formazione e non mette nelle medesime condizioni di qualità l'intero panorama dello Stato. Allora, va rimessa mano in questo ambito (dagli OSS, agli OSA, ai pedagoghi, agli psicologi

parlamentare, guadagni non solo nello spirito di risposta alle esigenze dei cittadini trasferite attraverso i propri parlamentari, ma guadagni moltissimo in questo sistema salute, riconoscendo tanto sforzo, tanto impegno ed una storia lunghissima di professionalità come finalmente facciamo in quest'Aula.

di alcuni militari. Molto brevemente, desidero poi informare l'Aula che è morto il signor Leone Massa. Molti di noi lo ricorderanno, perché è stato per tanti anni presidente dell'associazione degli imprenditori attivi in Libia e cacciati da Gheddafi 35 anni or sono. Purtroppo Leone Massa, malgrado fosse quotidianamente qui fuori, in Transatlantico, a insistere perché il Governo si assumesse una responsabilità relativamente a quei cittadini italiani (perché stiamo parlando di cittadini e imprenditori italiani maltrattati da Gheddafi), non ha visto coronare il suo sogno, cioè che, finalmente, venisse venisse prima l'amicizia con gli italiani e poi, eventualmente, anche quella, non con il popolo libico (ahinoi), ma con il dittatore Gheddafi. Dico ciò perché l'Italia ha scongelato due miliardi e mezzo di fondi libici investiti in Italia, che andranno al Consiglio nazionale transitorio libico. Ebbene, occorre trovare il modo, all'interno di questa ingentissima cifra, di recuperare quelli che sono, a questo punto, pochi spiccioli, in onore della memoria e dell'impegno di Leone Massa (al quale vanno i nostri più affettuosi ricordi e che, sicuramente, grazie a Radio Radicale, anche in Paradiso, dove sicuramente si trova, ci sta ascoltando), ma anche per andare incontro alle richieste di migliaia di italiani. Siamo riusciti, in qualche modo, a fare tutte le capriole possibili nei rapporti con la Libia. Ebbene, l'ultima giravolta utile è quella di prendere in considerazione le richieste sia dei cittadini italiani che degli imprenditori cacciati dalla Libia, trovando quelle poche centinaia di migliaia di euro (o milioni, visto che sono passati anni e sono maturati degli interessi) per recuperare, molto lentamente e veramente in «zona Cesarini», come si dice in gergo calcistico, un minimo di reputazione di fronte a noi stessi

ha emesso un'importante decisione con la sentenza n. 5032, chiudendo definitivamente la partita tra la Provincia di Pisa, CREDIOP e DEPFA, per i derivati avariati, vera e propria finanza criminale, criminale, appioppati ad oltre 500 enti locali per un valore nozionale di 52,2 miliardi di euro,

offrendo la possibilità ai contraenti (gli enti locali) dell'annullamento in autotutela davanti al giudice italiano, non già alle Corti inglesi cui si erano rivolte tali banche. Voglio ricordare ancora una volta i derivati avariati di Unicredit e di altre banche italiane ed estere, che hanno condotto al dissesto finanziario imprese solide, costrette a stipulare contratti capestro

ingegnerizzati, importati in Italia dal mondo anglosassone, i cui algoritmi offrivano possibilità alle banche di guadagnare il 90 per cento e ai contraenti di perdere sempre. Le grandi banche italiane non hanno resistito ai lauti profitti consentiti dai derivati *over the counter* fuori da mercati regolamentati) di copertura contro il rialzo dei tassi di interesse venduti a enti territoriali, imprese, società finanziarie che, secondo gli ultimi dati disponibili della Banca d'Italia al 31 dicembre 2010, registravano perdite - lo ripeto - del valore nozionale di 52,2 miliardi di euro. I derivati miliardi di euro. I derivati tossici hanno intossicato la vita a migliaia di imprese, enti locali e società finanziarie, che non sono riuscite più a far fronte alle rate crescenti da pagare. Continuerò, signor Presidente, a denunciare le malefatte di una finanza di carta che ha divorato l'economia reale, confidando che alcuni banchieri senza scrupoli, che hanno appioppato tali derivati truffaldini ad imprenditori ed enti locali, invece di essere candidati al ruolo di salvatori della Patria,

a persone che poi si lamentano perché pagano 8 euro il pasto al ristorante del Senato è molto umiliante, e che la classe dirigente che fa una simile è abbastanza miserrima.

Credo che dei servitori dello Stato, non dico al pari nostro, perché forse loro sono più servitori di noi, non si possano permettere di delegittimare un'istituzione come il Senato e dire che possono tirare i lacrimogeni in Senato. Normalmente si dice che la prima gallina che canta è quella che ha fatto l'uovo. Tengo a precisare, forse per quei pochi che avranno modo di seguire il mio intervento anche nella televisione interna, che non mi sento certo sfiorato da queste robe. Ho fatto il carabiniere, vengo da una famiglia molto povera, ma nobile d'animo, non ho mai gestito un euro strano in vita mia: non mi faccio mica dire da questi fenomeni quello che dicono! Se vogliono lanciare i lacrimogeni e vogliono che noi parlamentari... Mettiamo un attimo da parte

Mi meraviglia che nel Comitato elettorale ci dovrebbero essere delle persone sagge, come Sartori che fa il politologo. Se lui pensa che noi siamo dei maiali o che chi fa il parlamentare è un maiale credo che non vada proprio bene. Concludo dicendo, caro Presidente, che siamo partiti dal ritiro delle tessere delle autostrade e delle